Onorevoli colleghi, come già comunicato per le vie brevi ai Gruppi nella giornata di ieri, avverto che oggi, alle ore 19, il Ministro dell'interno renderà un'informativa al Senato sull'aggressione subita dal Presidente del Consiglio dei ministri a Milano.

*relatore*. Signora Presidente, il disegno di legge in esame, dopo il passaggio alla Camera dei deputati, pur essendo stato modificato in numerosi punti, non ha perso l'ispirazione di fondo ricevuta durante l'esame effettuato dal Senato in prima lettura. Giova dare conto comunque, di seguito, delle principali novità introdotte dalla Camera dei deputati, tralasciando, per brevità, tutte le numerose modifiche di semplice chiarimento o coordinamento interno. È stata modificata in alcune parti la delega prevista all'articolo 2, in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, ivi prevedendosi una serie di modifiche ai contenuti tecnici e procedurali concernenti l'avvio della riforma del sistema contabile secondo i canoni dell'uniformazione per tutti i comparti e settori della pubblica amministrazione. La scelta di fondo operata dalla Camera è stata quella di rinviare alla legge 5 maggio 2009, n. 42, (la legge sul federalismo fiscale), per la parte relativa ai criteri e principi di armonizzazione delle Regioni e degli enti locali, lasciando il resto al presente testo. Va ricordato peraltro che nel corso del dibattito è stato osservato che il testo del Senato sul punto aveva espresso in qualche modo una posizione centralistica. Probabilmente, chi ha manifestato un tale orientamento non ha tenuto in debita considerazione il fatto che quel testo già prevedeva l'intesa della Conferenza Stato-Regioni sugli schemi dei decreti legislativi della riforma in materia di armonizzazione dei bilanci. sempre il testo approvato in prima lettura conteneva diverse previsioni in tema di condivisione delle decisioni di finanza pubblica tra i vari livelli istituzionali per quanto riguarda il coinvolgimento delle autonomie nel processo deliberativo di cui alla legge di stabilità. Un'attenta lettura della normativa pertanto avrebbe portato ad esprimere una valutazione diversa sul punto del coinvolgimento delle autonomie. Sul tema degli strumenti informativi a supporto della decisione parlamentare è da segnalare che un'altra modifica è stata la soppressione della Commissione parlamentare per la trasparenza e l'informazione nel campo della finanza pubblica, per ricondurre il processo di verifica e controllo nell'ambito della sede delle Commissioni bilancio, che dovrebbero agire su questo versante di comune accordo. Sotto questo aspetto il dibattito in Commissione è stato particolarmente concentrato su quale modulo organizzativo sia più adatto per una riflessione non episodica anzitutto sui criteri usati per l'elaborazione delle previsioni del Governo. Alla maggioranza è sembrato che la soluzione della Camera non escluda un esame di tali aspetti, rimesso all'interno delle due Commissioni bilancio, eventualmente in sede congiunta. Sempre sotto il profilo del collegamento con la legge sul federalismo, sul federalismo, è stato deciso dalla Camera che, a livello normativo, è la nuova legge di stabilità ad occuparsi del patto di stabilità interno, mentre del patto di convergenza si può occupare anche un apposito provvedimento collegato, oltre che naturalmente la stessa legge di stabilità. Va sottolineato con forza il dato istituzionale di fondo di tale assetto, per l'estrema rilevanza delle materie ivi richiamate. Va espresso dunque compiacimento per il fatto che attraverso un'opportuna modifica della richiamata legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale sia stata ricondotta all'ambito di competenza della legge di stabilità la complessiva decisione sui saldi, sul debito e sulla pressione fiscale complessiva, con tutte le garanzie e le tutele previste in ordine alla collaborazione delle Regioni e delle autonomie alla definizione di tali obiettivi complessivi, secondo un quadro già pensato in prima lettura ma che poi non ha trovato sufficiente esplicitazione normativa. Sulle implicazioni di una tale decisione mi soffermerò alla fine della presente relazione. Per quanto concerne poi i contenuti della manovra di cui all'articolo 11 (nuova legge di stabilità), va segnalato il sostanziale ripristino dell'articolazione tabellare in essere, che infatti, dalla iniziale previsione di integrazione e semplificazione, ritorna alla indicazione separata delle tabelle C, E ed F, quest'ultima integrata dei contenuti della precedente tabella D. Si è stabilito poi che il disegno di legge di stabilità debba contenere, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali della manovra sui saldi di finanza pubblica. È stato altresì previsto dalla Camera che nei tre esercizi finanziari successivi alla approvazione del disegno di legge, i Ministri competenti presentino al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione dei relativi programmi di spesa e sul loro grado di avanzamento, prevedendo altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze possa disporre il mantenimento di residui per spese in conto capitale anche in deroga ai termini previsti dalla normativa di contabilità. Un'altra questione che va sottolineata è la sistemazione che la Camera ha operato per quanto riguarda il contenuto e la tempistica dei provvedimenti collegati. Già l'attuale legge 5 agosto 1978, n. 468, ribadita dal testo approvato dal Senato del presente disegno di legge, staccava, anche sotto il profilo del termine della presentazione dei relativi atti parlamentari, la figura del «collegato» dalla sessione di bilancio: la Camera ha ulteriormente accentuato questo distacco spostando il termine di presentazione dei «collegati» al mese di febbraio dell'esercizio successivo e prevedendo che la funzione normativa di sviluppo, non più tipica della nuova legge di stabilità, venga appunto convogliata nel provvedimento collegato *ad hoc*. Ne risulta pertanto un disegno complessivo che è bene sia chiaro nei suoi aspetti istituzionali di fondo - secondo cui al netto dell'eventuale manovra di sviluppo contenuta negli stanziamenti di bilancio e nella legge di stabilità per la parte relativa alle tabelle, tutta la componente normativa della politica di bilancio (norme sia di sviluppo che di carattere ordinamentale e organizzatorio) viene istituzionalmente concentrata ora nella figura del provvedimento collegato, di cui rimane il richiamo necessario nel nuovo DPEF, ossia nella Decisione di finanza pubblica. si è provveduto alla separata indicazione, con la creazione di un apposito articolo della delega, per il passaggio al criterio della cassa inizialmente contenuta in una lettera dell'articolo 43. dei criteri di configurazione dei bilanci pubblici si ricorderà che nel corso della prima lettura sono stati approfonditi i complessi e in parte irrisolti problemi connessi alla estendibilità o meno a tali bilanci della contabilità di tipo civilistico-patrimoniale: l'esito di tale problematicità era stata l'accentuazione nel testo del carattere sperimentale del passaggio a tale tipo di contabilità. La Camera ha risolto in modo *tranchant* il problema, sia pure nell'ambito di una implementazione che durerà qualche tempo, trattandosi di deleghe. In definitiva, ribadendo quanto affermato in premessa, va dunque osservato che il testo in esame, sia pure corredato di ulteriori numerose precisazioni, conserva l'ispirazione di fondo che già lo caratterizzava all'atto dell'approvazione avvenuta in prima lettura. Come avvenuto in occasione dell'approvazione della legge sul federalismo fiscale, anche in quel caso avvenuta in prima lettura da parte del Senato, è possibile peraltro dare un giudizio più che positivo sulla convergenza anche dell'altro ramo del Parlamento sulle scelte fondamentali inerenti la configurazione nuova che andrà a caratterizzare gli strumenti di governo della finanza pubblica in Italia. Restano comunque alcuni aspetti che necessiterebbero di un chiarimento. Tra questi si segnala, anzitutto, la previsione contenuta nell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, appena convertito, con modificazioni, dalla legge legge 20 novembre 2009, n. 166, della trasmissione da parte di Regioni e Province autonome alla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo dei dati contabili risultanti dai rendiconti secondo lo schema contabile allegato al decreto stesso, materia, questa, espunta dal presente testo. Va da sé che la sede dove la questione dovrebbe trovare la propria regolamentazione è appunto la legge che ci apprestiamo a varare. In merito il Governo ha fatto presente in Commissione che la soluzione legislativa assunta non altera comunque la costruzione e la logica complessiva del disegno di legge in esame. Un altro dei problemi è la reintroduzione della copertura degli oneri correnti della legge finanziaria mediante il ricorso al miglioramento del risparmio pubblico, il che ha comportato il venir meno di un'altra innovazione fissata dal testo del Senato, ossia la facoltatività della presentazione facoltatività della presentazione da parte del Governo del disegno di legge di assestamento. Si tratta di un complesso di questioni su cui il Senato aveva riflettuto molto in prima lettura, propendendo per una linea più moderna che lasciasse complessivamente il Governo libero di impostare la politica di bilancio, spostando dunque il limite giuridico ai saldi complessivi. Con la soluzione pervenutaci rimane l'obbligo di copertura della legge di stabilità, nonostante esso sia da tempo scaduto ad un livello abbastanza formale proprio per l'assenza di meccanismi che consentano un esame penetrante della congruità delle poste del bilancio a legislazione vigente, il che costituisce però la premessa per la effettività di un obbligo di copertura costruito in tal modo. Il compito che abbiamo davanti non è semplice, pertanto, e la questione non sembra trovare al momento una soluzione soddisfacente, riproponendosi così un assetto ordinamentale che si è dimostrato nel tempo abbastanza privo di sostanza. Tra l'altro, la formulazione della Camera circa il riferimento al carattere positivo del risparmio pubblico, da garantire comunque, dovrebbe essere inteso nel senso che, nell'ipotesi che il saldo corrente dell'assestamento abbia un segno negativo mentre quello del bilancio di previsione presenti un carattere positivo, il margine utilizzabile a copertura dovrebbe estendersi fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della possibilità di utilizzare la parte negativa. Di questo ci sono stati esempi nel passato e quindi questa precisazione nella relazione. Su tale complesso di problemi, sempre nel dibattito in Commissione, il Governo ha fatto presente che la soluzione della Camera può rappresentare un utile strumento per evitare o ridimensionare gli eventuali effetti di ricomposizione della spesa dal conto capitale a parte corrente derivanti da emendamenti approvati dal Parlamento, potenzialmente possibili con il testo approvato dal Senato in prima lettura. In merito poi alla interpretazione fornita sui limiti di utilizzo del risparmio pubblico, il Governo ha convenuto sulla interpretazione che esso sia utilizzabile fino all'azzeramento del margine, con esclusione quindi della parte negativa, nel caso in cui il miglioramento sia riferito al passaggio da un valore negativo (indicato nell'assestamento) ad uno positivo (nel bilancio di previsione). In definitiva, appare chiaro sul punto che deve essere rafforzato l'impegno in tutte le sedi per una verifica dei criteri di costruzione dei tendenziali, in maniera che si eviti il rischio di una loro conformazione anche in vista del reperimento dei mezzi aggiuntivi di copertura. Altra questione su cui probabilmente occorrerà ritornare è il fatto che per la legge di stabilità sia stato previsto un divieto di norme localistiche e microsettoriali, il che appare abbastanza incongruo se si considera che il provvedimento ha perso la propria componente normativa di sviluppo, con il risultato dunque che al momento non sarebbe possibile prevedere un contenimento ovvero una variazione di aliquote settoriale o localistica. Sul punto, nel dibattito in Commissione, il Governo ha ritenuto che la problematica non sussista, posto che la disposizione (articolo 11, comma 3) non parla genericamente di norme, ma di interventi. In questo senso, la limitazione riguarderebbe esclusivamente le misure di carattere espansivo. Anche in questo caso mi è parso opportuno reintrodurre questa problematica all'interno della relazione, proprio perché nel dibattito parlamentare questi concetti siano assolutamente chiariti. Un chiarimento va fatto poi per quanto riguarda la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 40, che, nel prevedere come criterio di delega la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire, va ovviamente interpretata nel senso che si tratta solo di organizzare, se si modifica il contenuto dei programmi, il relativo gruppo di leggi che insistono sul medesimo programma. Va dunque esclusa qualsiasi ipotesi che attraverso la delega in questione si possa in via amministrativa modificare la legislazione di merito. Anche su questo punto il Governo ha concordato sulla considerazione che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione vada interpretata nel senso di una riorganizzazione del contenuto dei programmi, escludendo qualunque ipotesi che preveda modifiche della legislazione con atti di carattere amministrativo. In linea generale, il dibattito in Commissione è stato particolarmente ricco e approfondito. Per alcuni aspetti se ne è fatto già cenno. Vale la pena qui riprendere brevemente altri temi tra i più rilevanti. Per quanto riguarda i rilievi mossi in relazione all'articolo 8, in tema di patto di stabilità interno, è stato anzitutto fatto presente che le critiche alle modifiche della Camera devono essere intese come un auspicio perché le norme in materia non vengano ridiscusse e ridisegnate ogni anno nella legge di stabilità: questo è lo spirito delle modifiche della Camera. Per quanto riguarda l'argomento secondo cui all'articolo 17, comma 4, sarebbe stato introdotto in via surrettizia l'obbligo di copertura sui tre saldi, si ricorda che comunque ciò è limitato ai casi in cui è prevista la relazione tecnica, il che più o meno corrisponde più o meno corrisponde a quanto già avviene. Non c'è stata dunque nessuna surrettizia introduzione dell'obbligo generalizzato di prevedere la copertura sui tre saldi: vorrei che questo fosse ben chiaro, perché sul punto il dibattito in Commissione è stato particolarmente vivace. Si tratta peraltro di una questione che attiene alle modalità di svolgimento dell'iniziativa legislativa di ciascun parlamentare e quindi della massima rilevanza politica ed istituzionale. Ciò introduce all'altro argomento circa la soppressione dell'obbligo della relazione tecnica per quanto riguarda il relatore: poiché la questione rimane rimessa ai Regolamenti parlamentari sarà in questa sede che eventualmente si provvederà al riguardo. Sempre per quanto riguarda l'articolo 17, in ordine alla soppressione delle parole «o non ricorrenti» dalla lettera ossia la impossibilità di usare a copertura entrate non ricorrenti, anche qui l'auspicio, in sintesi, è che i vincoli crescenti sull'indebitamento netto producano in sostanza, nei fatti, un obbligo di copertura aderente allo spirito della norma del Senato. Per quanto riguarda il quesito posto, a proposito del contenuto della legge di stabilità, circa il divieto di introdurre norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, fatto salvo quanto previsto in tema di patto di stabilità interno in tema di patto di convergenza, sembrerebbe potersi concludere nel senso che sono ammissibili norme di carattere ordinamentale od organizzatorio quando esse siano connesse al patto di stabilità interno o al patto di convergenza e, quindi, servano a regolare entrambe le materie, a prescindere dall'effetto sui saldi. Si tratta di un'interpretazione che *melius* *re* *perpensa* nasce dal fatto che con apposita norma si è voluto caratterizzare il «collegato» come la sede per prevedere questo tipo di norme, a prescindere dal segno dell'intervento. Vorrà dire che, se ci saranno effetti positivi, essi, in quanto non spesi, verranno acquisiti ai saldi. Rimane dunque la linea del non appesantimento della legge di stabilità. Per quanto riguarda poi la possibilità, in riferimento all'articolo 21, comma 2, che il coordinamento con il secondo livello COFOG (*Classification per quanto riguarda l'articolo 17, relativo alla cassa, in effetti la nuova versione della norma implica maggiori cautele rispetto ad un passaggio effettivo rispetto ad un sistema di cassa: trattandosi comunque di una delega, anche in questo caso l'invito al Governo è di pervenire ad una proposta con i decreti delegati che sciolga i vari dubbi interpretativi che la norma comporta. A tal riguardo, mi sia permesso aggiungere la particolare cautela che il Governo dovrà porre nel dare attuazione al numero 2), della lettera *b)*, del comma 2 dell'articolo 40, a proposito del quale si deve evitare, come riusciva a fare la versione approvata dal Senato, la proliferazione dei centri di responsabilità amministrativa per assicurarne la corrispondenza con ciascun programma di spesa: in caso contrario, la normativa rischierebbe di comportare oneri, pericolo che il testo del Senato - ribadisco - voleva evitare. Per quanto riguarda poi le due criticità relative alla necessità di rendere più marcato l'obiettivo della pressione fiscale e ad un'esigenza di avere una maggiore documentazione da parte del Governo nella materia della lotta all'evasione, ricordo che, per quanto concerne il primo punto, la questione è stata a lungo dibattuta anche in prima lettura e l'orientamento, almeno della larga maggioranza che ha votato il testo sia al Senato che alla Camera, è stato di evitare di far assumere a tale obiettivo una valenza più stringente. La questione è complessa, ma le perplessità si possono riassumere nel fatto che la pressione fiscale dipende in larga parte da eventi sui quali la decisione politica può

e del tessuto produttivo. Per quanto riguarda il secondo punto, ossia l'esigenza di una relazione più dettagliata sulla lotta all'evasione, il testo sia al Senato che alla Camera è stato robustamente corroborato di indicazioni che il Governo deve fornire per quanto riguarda le agevolazioni fiscali varate con i relativi effetti. Questo non esclude che il tutto possa essere migliorato con relazioni che si possono richiedere di volta in volta, a seconda delle esigenze e degli andamenti. Anche in questo caso la questione potrà essere oggetto di un ordine del giorno. Il complesso delle considerazioni formulate mi porta ad auspicare, in definitiva, un'approvazione senza ulteriori modifiche del testo al nostro esame. Evidente è la circostanza secondo cui l'impegno riformatore del Parlamento in questa materia non si conclude in questa sede. Il complessivo testo all'esame prevede infatti un'articolata sequenza procedimentale di attuazione, sulla quale il Parlamento sarà chiamato nei prossimi mesi, a rinnovare il proprio impegno e la propria costante attenzione. Prima di concludere, vorrei far presente un punto di particolare rilievo. Il recente dibattito in Senato sulle mozioni in materia costituzionale mi induce ad una riflessione, che poi avrà un seguito nel confronto con le forze politiche e con il Governo quando si dovesse pervenire all'esame dei testi di riforma della Costituzione. Alludo al fatto che il testo in esame sottolinea con forza in vari punti un'articolazione della manovra (e ancor prima dei quadri tendenziali e programmatici) che metta in rilievo la suddivisione degli obiettivi per sottosettori istituzionali (Stato, Regioni, enti locali, eccetera). Ciò è dovuto non solo ad esigenze oggettive, come dimostra la analoga configurazione da tempo dei vari Programmi di stabilità quali vengono inviati a Bruxelles, ma anche al fatto che, se in futuro il Senato dovesse essere strutturato sulla base di un assetto federale e l'impianto istituzionale effettivo del Paese sarà veramente improntato a tale ultimo principio, come tutti auspichiamo, è del tutto ovvio che la decisione-quadro sulla suddivisione preliminare della manovra (ed anche di quelle espansive in riferimento ai provvedimenti collegati) non potrà che essere assunta in una sede, appunto, il Senato federale, espressione di tutti i sottosettori, ossia di tutti i livelli politici ed istituzionali che vanno a comporre l'aggregato pubblica amministrazione. Spetterà poi al complesso esecutivo-legislativo di ogni sottosettore, compreso quello a livello statale, decidere come regolare la quota di saldo complessivo spettante al livello di appartenenza, dopo che è stata assunta la decisione-quadro nel suo complesso. Era questo il disegno della legge di riforma del 2005 (poi non confermato dal *referendum*) sulla base delle indicazioni emerse da parte di tutte le componenti del centro-destra ed è questo il disegno riformatore più logico e coerente che dovrà essere ripreso quando si ridiscuterà

negli Stati Uniti d'America da settimane infuria una violenta polemica tra repubblicani e democratici (ma anche dentro ognuno di questi due partiti) sulla riforma sanitaria. I sostenitori della riforma e quanti la avversano organizzano manifestazioni, petizioni, capillari mobilitazioni di piazza in ogni città e villaggio degli Stati Uniti. Entrambi gli schieramenti fanno ricorso all'intervento pubblico dei migliori economisti ed esperti; sui giornali e nelle televisioni scrivono e parlano premi Nobel e credibili aspiranti al premio Nobel. È uno scontro duro senza esclusione di colpi, ma nessuno dei combattenti contesta le analisi del *Congressional Budget Office* circa i costi della riforma prevista, il suo impatto sui conti pubblici nell'immediato e nei prossimi dieci anni. Con le sue analisi il CBO ha vistosamente corretto quelle di Peter Orszag, l'uomo dei numeri del presidente Obama, che aveva presentato stime diverse sull'impatto finanziario della riforma. I numeri, dunque, sono quelli del CBO. Sulla loro interpretazione, sui giudizi da trarne è aperto il conflitto politico: non sull'attendibilità dei numeri. Ecco ciò che ci manca, signor Vice Ministro, signori colleghi: il Servizio del bilancio del Parlamento italiano nel quale fondere le ottime energie, risorse culturali, scientifiche e tecniche già oggi presenti nei due Servizi del bilancio di Camera e Senato, da considerare la base da cui partire per un grande rafforzamento, capace di colmare - questo è il punto cruciale della discussione che noi stiamo facendo facendo - l'insopportabile divario di conoscenza, informazione e capacità di analisi tecnica che oggi separa il Parlamento dal Governo. un divario, una asimmetria informativa che - lo dico a quanti tra noi e nel sistema delle autonomie regionali e locali pensano che questi siano problemi per iniziati, sostanzialmente trascurabili per chi si occupa di politica diventeranno nei prossimi mesi ed anni letteralmente insostenibili quando si dovrà passare all'attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale. Allora tutti scopriranno che il Governo, o meglio una struttura del Governo interna al Ministero dell'economia - la Ragioneria generale dello Stato - detiene il monopolio dell'informazione. A quel punto i dati - ecco il danno che deriverà dal problema che sto affrontando e dalle soluzioni che la Camera ha improvvidamente adottato su questo punto - ripeto, i dati, non le scelte politiche, diventeranno oggetto di scontro politico e tutto diventerà più difficile per l'attuazione della legge sul federalismo fiscale in primo luogo. Ecco perché qui al Senato, insieme - maggioranza, opposizione e Governo - avevamo scelto di aggredire il problema in radice: struttura unica di supporto tecnico del Parlamento (articolo 7 del testo approvato dal Senato); accesso diretto, automatico e garantito, di questa struttura a tutte le banche dati rilevanti per il monitoraggio della finanza pubblica; Commissione bicamerale vocata ad occuparsi non, come recita l'attuale testo della legge modificato alla Camera, del controllo degli andamenti di finanza pubblica, perché di questo degli andamenti di finanza pubblica, perché di questo ovviamente si occupano le Commissioni bilancio permanenti e non c'è bisogno di fare nessuna Commissione bicamerale, ma di sovrintendere a tutto il processo di iniezione di trasparenza nel sistema, a partire questo è il nodo cruciale - dalla conoscenza delle metodologie usate per la costruzione degli andamenti tendenziali di finanza pubblica a legislazione vigente vigente con «evidenziazione delle basi conoscitive necessarie per la loro verifica», come recitava il testo di legge approvato dal Senato e come purtroppo non recita più la legge uscita dalla Camera. Questo infatti è il nodo da sciogliere: se noi vogliamo davvero concentrare l'attenzione non sugli interventi ai margini, come facciamo da anni ormai, sulle variazioni minimali della spesa pubblica e delle politiche di prelievo che la finanziano, ma sull'intera spesa pubblica, sui risultati conseguiti attraverso quella spesa, noi Parlamento dobbiamo prima di tutto capire attraverso quali metodologie - proprio così - si costruisce il documento base di tutta la decisione di bilancio che, com'è noto, è il bilancio tendenziale a legislazione vigente. Se noi non conosciamo le metodologie attraverso le quali si costruisce questo documento tutto il resto della decisione di bilancio lo conduciamo al buio. Questa è la verità. Prima ancora dobbiamo conoscere le metodologie attraverso le quali viene costruito il quadro tendenziale a legislazione vigente del Documento di programmazione economico-finanziaria che è la base per costruire il bilancio a legislazione vigente; quel DPEF che domani, sulla base di questa legge, si chiamerà Decisione di finanza pubblica. Per questo la decisione della Camera, assunta all'unanimità, all'unanimità, non di emendare ma di abrogare, eliminare sia la struttura tecnica sia la Commissione bicamerale per la trasparenza, sottoponendo poi il collegamento del Parlamento alle banche dati del Governo ad improbabili apposite intese da fare successivamente, e che naturalmente non si faranno mai, è una decisione assai grave, tale da giustificare da sola un mutamento del nostro giudizio su questa legge. Se la maggioranza e il Governo non accetteranno di modificare il testo su questo punto noi non potremo confermare il voto favorevole che abbiamo dato in prima lettura. Perché la Camera ha preso una decisione così negativa? La mia personale opinione è che cercheremmo invano la risposta nell'esame dell'orientamento e delle posizioni dei Gruppi politici. No: ad imporsi sono state le posizioni conservatrici dell'unico grande, qualificato apparato burocratico che possiede oggi le conoscenze, le informazioni e le competenze tecnico-scientifiche necessarie per ergersi a *dominus* dell'intero campo: la Ragioneria generale dello Stato. Una struttura che ha potuto contare, a questo fine, sulle resistenze conservatrici delle burocrazie parlamentari, in specie quelle della Camera dei deputati. Perché, colleghi, dovremmo piegare la testa di fronte a questo conservatorismo, che non è né di destra né di sinistra, ma è conservatorismo e basta? Tra qualche tempo, signora Presidente, comincerà a lavorare la Commissione bicamerale per l'esame dei decreti legislativi delegati sul federalismo fiscale.

dei costi standard, compiendo così scelte destinate ad incidere profondamente nella carne viva del Paese? La Commissione chiederà improbabili, estemporanei e magari anche costosi aiuti a questo o quel dipartimento universitario, che per la prima volta affronterà il tema, oppure, come io temo, prenderà per buoni temo, prenderà per buoni i dati forniti dal Governo, senza che quest'ultimo abbia l'obbligo di chiarire (torno al tema) quali siano le metodologie di raccolta e elaborazione di quei dati?

l'autonomia tecnico-scientifica e di conoscenza dell'organo di controllo rispetto al controllato, cioè del Parlamento rispetto al Governo. Per questo motivo insisto, rivolgendomi ai colleghi della maggioranza

ma la capacità della nuova legge di contabilità di corrispondere alle esigenze che nascono dalla fase attraversata dal Paese. Ciò è tanto più vero, colleghi della Lega Nord e del PdL, se prendiamo sul serio, come ha fatto adesso il relatore con un atteggiamento che io ho apprezzato, l'ipotesi di riforma del Parlamento che tutti diciamo di condividere: una sola Camera politica e il Senato federale. del provvedimento in esame, se un Parlamento così riformato, Camera politica e Senato federale, possa essere privo di una sede tecnica autorevolissima e unitaria di analisi sui dati di finanza pubblica. È accettabile, colleghi della Lega, che in uno Stato federale il Governo centrale possieda in questo campo un monopolio indiscusso e indiscutibile? Su altri rilevantissimi aspetti delle modifiche introdotte dalla Camera interverrò in sede di illustrazione degli emendamenti. In questa sede voglio solo richiamare due aspetti che io considero molto rilevanti. Il primo è la la modificazione, ma la soppressione - dei due commi dell'articolo 8, con i quali il disegno di legge del Senato disponeva nuove regole in tema di Patto di stabilità interno (Patto di stabilità interno, collega Garavaglia).

dal Senato, accogliendo un emendamento del gruppo del Partito Democratico, era rivolto (lo dico rifacendomi alla famosa frase del presidente Prodi, allora presidente della Commissione europea) a rendere meno stupido il Patto di stabilità interno. Per la spesa in conto capitale, infatti, quel testo introduceva la possibilità che i Comuni potessero, alla dimensione regionale e fermo restando l'obiettivo da conseguire, fissato nel Patto di stabilità interno e incorporato per gli obiettivi quantitativi e numerici nella legge di stabilità di ogni anno, scambiarsi reciprocamente i diritti di indebitamento. Era una regola che, in ogni Regione, avrebbe favorito, ogni anno, il raggiungimento del *top* delle scelte d'investimento degli enti locali, senza compromettere minimamente il rispetto del Patto di stabilità nazionale. Si poteva modificare, si poteva trovare una regola diversa, migliore di questa. La scelta di abrogare adottata dalla maggioranza della Camera la trovo invece inutilmente penalizzante e, se mi è consentito, un po' stupida; che sia stata presa con il consenso del mondo delle autonomie locali ci dice solo che anche in quel caso forse ci sono rapporti di potere da mettere radicalmente in discussione. Sul secondo punto il problema fondamentale dei Paesi ad elevatissimo livello di debito pubblico (nel novero dei quali purtroppo rientriamo, com'è noto) è quello di dare profondità temporale alle decisioni di finanza pubblica, perché con la gestione anno per anno non si riesce mai ad affrontare strutturalmente il problema del rientro dal debito pubblico, così da dotarsi di una credibile strategia di medio-lungo periodo, una credibile strategia di medio-lungo periodo, l'unica che può avere successo in contesti caratterizzati da elevatissimo livello del volume globale del debito. Per fare questo è indispensabile interrompere la spirale che considera la spesa (sembra di tornare ai primi anni Settanta ed al dibattito sindacale) una variabile indipendente e la pressione fiscale la variabile ancella, che deve inseguire la prima (ve lo ricordate il salario variabile indipendente?). La definizione degli obiettivi in termini di solo saldo è figlia di questa cattiva pratica, per la ragione ovvia che l'obiettivo di saldo si può raggiungere sia riducendo la spesa sia, naturalmente, aumentando le entrate; la strada che seguiamo sistematicamente, considerando la spesa una variabile indipendente, è quella dell'aumento delle entrate: la pressione fiscale che insegue e si adegua all'aumento della spesa fuori controllo. Di qui la scelta che avevamo fatto al Senato di un'indicazione distinta degli obiettivi di spesa primaria e di pressione fiscale, in maniera tale che distintamente si potessero compiere scelte politiche in rapporto ai due obiettivi programmatici. Certo, era solo a fini conoscitivi, l'obiettivo impegnativo rimaneva quello del saldo, ma quei fini conoscitivi sono la premessa per poter poi impostare anche obiettivi politicamente più impegnativi. Poco male, dirà qualcuno, in fondo tutto ciò era previsto solo a fini conoscitivi; non sono d'accordo e, se guardo a questa scelta alla luce di quella operata della Camera sull'articolo 17 (ex articolo 18 del testo del Senato) per consentire la copertura - attenzione colleghi - con entrate non ricorrenti di oneri correnti (perché il testo del Senato è stato modificato alla Camera per consentire che oneri correnti siano coperti da entrate non ricorrenti), guarda caso, quest'anno c'è proprio un chiaro esempio di tale scelta, perché le entrate da scudo fiscale sono entrate non ricorrenti. Il testo del Senato invece questa soluzione la vietava. Il testo della Camera elimina le paroline "non ricorrenti", con il risultato che si possono coprire oneri correnti con entrate non ricorrenti. E se poi guardo a questa norma di cui mi sto occupando alla luce delle modifiche apportate all'articolo 11, comma 6, per consentire di usare il miglioramento del risparmio pubblico - ne ha parlato il relatore a copertura di nuovi oneri recati dalla legge finanziaria, che diventerà legge di stabilità, posso constatare che anche questa possibilità il testo del Senato non l'aveva prevista, non perché si era dimenticato di prevederla, ma perché non voleva prevederla, poiché voleva vietare

in un Paese che ha un volume globale del debito come il nostro, se c'è un miglioramento del risparmio pubblico cosa bisogna farne? Coprire nuovi oneri che nel frattempo si determinano con nuova spesa, oppure usare quel miglioramento del risparmio pubblico per far fronte al volume globale del debito troppo grande? Non c'è bisogno di essere

mi chiedo se questo insieme di scelte non nasconda un pericoloso cedimento lassista del Governo, coperto poi nel dibattito pubblico dalla retorica sul rigore finanziario che impedirebbe di fare scelte impegnative per affrontare la recessione. *(Applausi dai

di euro al mese, arrivando, come tutti sanno, a circa 1.801,6 miliardi di euro. La questione è proprio questa:

1.943,784 miliardi di euro, con un gravame pari a 32.936 euro per ogni cittadino, neonati compresi o, se si preferisce, di 92.561 euro per ogni nucleo familiare. Queste sono le cifre, questi sono i dati e su questo

su quelle spese che potrebbero essere comprimibili, perché poi la riforma della contabilità e della finanza deve avere la finalità di poter incidere anche sui rapporti tra Parlamento e Governo. A tal proposito, voglio ricordare - mi correggerà

concorrere alla definizione del ruolo delle Assemblee legislative nel sistema politico-istituzionale, per impedire che il Parlamento - a prescindere dai Governi e dalle maggioranze di tutti i colori - possa diventare mero esecutore di decisioni assunte assunte dall'Esecutivo, spesso senza alcun coinvolgimento nella delicata gestione della finanza pubblica. La necessità di una riforma della legge n. 468 del 1978 nasce dall'espansione del ruolo delle autonomie territoriali, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, dai vincoli imposti dall'Unione europea (il Patto di stabilità e di crescita e il conseguenziale Patto di stabilità interno), ma anche dalla riforma federalista con il relativo patto di convergenza quale strumento per realizzare l'obiettivo, per l'appunto, della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali. Con l'approvazione di questa riforma si delega il Governo ad adottare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni. revisione delle missioni in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi perseguiti con la spesa pubblica; revisione del numero e della struttura dei programmi in modo da assicurare un'univoca corrispondenza fra programma, risorse e strutture assegnate a ciascun Ministero l'affidamento di ciascun programma di spesa ad un unico centro di responsabilità amministrativa; revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e della relativa legislazione in coerenza con gli obiettivi da perseguire;

previsione che le nuove autorizzazioni legislative di spesa debbano essere formulate in termini di finanziamento di uno specifico programma di spesa; introduzione della programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato, nonché individuazione di metodologie comuni al fine di definire indicatori di *performance* semplici, misurabili e riferibili ai programmi di bilancio; introduzione di criteri e modalità per la fissazione di limiti per le spese rimodulabili del bilancio dello Stato. Tali limiti devono essere individuati in via di massima con la Decisione di finanza pubblica e successivamente devono essere adottati con la legge di bilancio, coerentemente con la programmazione triennale delle risorse. l'adozione, coerentemente con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri, in cui sono concordati gli obiettivi triennali e i tempi di conseguimento degli stessi; il riordino delle norme; l'accorpamento dei fondi di riserva e speciali; l'affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, a scopo conoscitivo e in via sperimentale, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale avente la funzione di verificare verificare i risultati conseguiti da parte delle amministrazioni, al fine di elaborare di conseguenza uno stato patrimoniale, un conto economico ed una nota integrativa, così come avviene per tutti i bilanci; la revisione del conto riassuntivo del Tesoro; la progressiva eliminazione, entro due anni, delle contabilità speciali o dei conti correnti di tesoreria; la previsione della possibilità di identificare contributi speciali, ed

per la cronaca, che al Presidente dell'ISTAT, in un momento in cui si tagliano gli stipendi, sono stati deliberati aumenti di stipendio del 330

giudizio abbastanza positivo; naturalmente non ci nascondiamo dietro un dito, perché questa riforma della legge di contabilità dello Stato, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 e della legge n. n. 42 del 2009, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, dovrebbe porsi l'obiettivo di delineare un riordino complessivo nella prospettiva della realizzazione di una contabilità della Repubblica, così come delineata dall'articolo 117 della Carta costituzionale. Questa disposizione, infatti, mentre assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni l'armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Anche gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere oggetto di intesa, da sancire in sede di Conferenza unificata.

finanza pubblica. Colleghi senatori, vice ministro Vegas, a distanza di circa otto anni dalla definizione della riforma del Titolo V della Costituzione, dopo l'approvazione nel maggio 2009 della legge delega sul federalismo fiscale, con questo disegno di legge di riforma della contabilità pubblica l'obiettivo di armonizzare i sistemi di finanza pubblica alla luce della recente riforma dell'amministrazione statale, in attesa dell'approvazione in sede parlamentare del cosiddetto codice delle autonomie cosiddetto codice delle autonomie varato a novembre dal Governo. Non è un momento neutrale nel complesso disegno governativo teso alla valorizzazione della funzione dello Stato quale motore

l'odierna legge di riforma. Il passaggio in Aula delle norme oggi in discussione non ha fatto perdere, come è stato rilevato nella relazione, l'ispirazione di fondo

Quali sono dunque i valori ai quali si ispirano le norme che stiamo esaminando? Innanzitutto, quelli della leggibilità di ogni scelta, che deve essere fatta all'interno di obiettivi progettuali chiari e nell'ambito di un'armonizzazione complessiva dell'azione complessiva dell'azione amministrativa, che non può procedere più al di fuori di un disegno unitario tra i vari livelli pubblici. Da qui discende la scelta politica di coinvolgere le amministrazioni locali nel Patto di stabilità: che Dio ce la mandi buona! Così il Governo potrà mettere in campo elementi premianti per chi meglio compie il proprio lavoro. Nel sistema di *governance* che si va prospettando sarà soprattutto necessaria la leale collaborazione tra i livelli di Governo, in modo da consentire il passaggio da una situazione di condizionamento reciproco di uno stretto coordinamento tra centro e periferia, con il superamento dello schema che ha spesso combinato le norme rigide imposte dall'alto con la mancanza di trasparenza e i vincoli di bilancio non rigidi per il sistema delle autonomie.

ed una omogeneizzazione dei criteri generali della finanza pubblica,che è una misura eccellente. dei rapporti tra centro e periferia che la riforma costituzionale ha delineato e l'ulteriore *input* che si attende dal combinato della delega sull'articolo 119 della Costituzione con il nuovo codice delle autonomie consentiranno miglioramenti di efficienza nel settore pubblico e maggiore comprensione da parte dei cittadini dei meriti e delle responsabilità (e questo finalmente, perché

La stessa cosa accadrà anche ai membri del Parlamento: finalmente, saremo in grado di leggere più agevolmente i conti pubblici e comprendere la portata delle scelte che l'amministrazione ad ogni livello farà. Siamo a buon punto nel lavoro di riforma in senso sempre più liberale, cioè attento alla modernità dell'uomo e della nostra macchina statale. condivido l'opinione del relatore, secondo cui l'impegno del Parlamento in questa materia non si conclude in questa sede: c'è ancora da lavorare e la riforma in senso federale dello Stato richiede infatti ulteriori miglioramenti della materia finanziaria e contabile. Penso tuttavia che il vero salto riformatore ci sarà quando i soggetti deputati a realizzare questo rinnovamento avranno assorbito realmente la nuova cultura che si sta inoculando nella burocrazia. Il principio di dover rendere conto ai cittadini utenti, agli elettori ed alle proprie comunità locali è di per sé un'innovazione rivoluzionaria rispetto ai pagamenti a piè di lista cui nella prima

ad ogni livello. A quest'ottica espressa nelle norme in esame va il mio voto favorevole e convinto. Vi ringrazio per l'attenzione. Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, quando abbiamo iniziato a discutere di questo argomento, vi erano con chiarezza due questioni di fronte a noi:

quanti soldi si prendono, dove e come si prendono e per fare che cosa; si tratta della base della nascita della democrazia parlamentare.

crisi globale che ha attraversato il nostro pianeta e che ci lascia un'eredità di interventi di carattere strutturale che vengono richiesti alla funzione pubblica. Per altro verso, vi era anche la consapevolezza che il bilancio dello Stato è parte di una più complessiva gestione dell'area pubblica: da un lato, è maggiormente vincolato rispetto al passato, per l'inserimento in un processo più ampio di equilibrio finanziario a livello europeo; dall'altro, è anche limitato dal crescere di una soggettività del sistema delle Regioni e delle amministrazioni. In senso proprio, si tratta anche di un bilancio dello Stato che assume una certa marginalità rispetto al più ampio recinto del conto consolidato della pubblica amministrazione, che diventa una grandezza molto più significativa anche nell'ambito delle politiche fiscali a livello europeo. La seconda questione consisteva nel regolamentare meglio il rapporto tra la funzione di governo e quella parlamentare, che ha subito una gravissima alterazione nel corso del tempo, modificando quel equilibrio bilanciato che era sotteso dall'articolo 81 della Costituzione. Ricordo ancora una volta che tra il 1995 e il 2002

nelle dichiarazioni, nelle interviste e nelle promesse anche di fronte all'opinione pubblica. Nella conduzione pratica, però, degli atti di governo non si è visto in nessun modo una convergenza: in attesa di

ho letto in questi giorni uno studio interessante che ha presentato il Servizio del bilancio del Senato in cui si dimostra che il 90 per cento degli oneri finanziari

sono derivanti da iniziative parlamentari. In queste due cifre c'è la gravità dell'alterazione di questo rapporto, confermata del resto anche dalla finanziaria di quest'anno,

ricordo, per misurare ancora una volta la forte separazione tra realtà e fatti, che la maggior parte dei proventi dello scudo fiscale va a finire in un fondo indifferenziato e globale presso la Presidenza del Consiglio, che rappresenta la negazione della trasparenza del bilancio e la negazione di quei principi che faticosamente si è cercato di scrivere in questo disegno di legge. Adesso ci troviamo di fronte ad un testo che ritorna dalla Camera con modifiche profonde, anche su parti decisive che erano state oggetto al Senato di un'azione convergente di maggioranza e opposizione. Penso che questo sia

Il giudizio sintetico che mi sentirei di esprimere è che, rispetto al testo licenziato dal Senato, le cose aggiunte vanno sostanzialmente bene: colmano in parte alcune lacune che l'opposizione, ma anche esponenti della maggioranza avevano evidenziato nel corso dell'esame al Senato. Sono le cose tolte, però, che vanno veramente male e che segnano, a mio avviso, un ripiegamento di notevole gravità rispetto all'ambizione di introdurre

con l'approvazione di queste norme si faranno dei passi in avanti: vi saranno una procedura più ordinata e trasparente, un miglioramento della base informativa nelle nelle procedure della sessione bilancio, la revisione della struttura di bilancio - con una più stretta corrispondenza tra programmi, risorse e strutture - che era stata uno dei motivi della scarsa efficacia della precedente riforma.

se non siamo in grado di mettere in discussione una modesta burocrazia parlamentare, l'altrettanto modesta ambizione delle due Commissioni

Questo è un problema che resta purtroppo irrisolto. Vi è poi il tema di un eccesso di centralizzazione del Tesoro in ogni decisione. decisione. Abbiamo visto dall'esperienza passata che per incidere sul serio nei meccanismi di spesa occorre anche una maggiore soggettività dei Ministeri di spesa,

conclusione, quando ormai trent'anni fa il ministro del Tesoro Beniamino Andreatta introdusse il cosiddetto divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro, attraverso cui la Banca d'Italia veniva liberata

degli interessi toccati, degli apparati burocratici e della difficoltà di aprire una fase totalmente nuova. Ci fu il coraggio della politica, ci fu la capacità di rompere le incrostazioni guardando al futuro. Dispiace che

Mi auguro che la fase sperimentale che comunque ci attende consenta, come dicevano gli antichi, di poter dire: «*crescit eundo*»; che nel percorso di attuazione, quando si toccheranno di nuovo i nodi irrisolti, quando si faranno i decreti attuativi, quando si dovranno affrontare le riforme costituzionali, si trovi quel coraggio che in questa occasione, ahimè, è mancato.

il Gruppo dell'Italia dei Valori ha piena consapevolezza che la riforma delle regole che governano la redazione e la presentazione dei conti pubblici, tra l'altro già più volte affrontate in passato a cadenza quasi decennale, è oggi diventata, al di là del dibattito politico che alterna tra i due rami del Parlamento momenti di enfasi e di criticità, e di criticità, una necessità non più rinviabile se viene però realmente affrontata nella nuova cornice, che è quella degli obblighi e dei vincoli dell'Unione europea e, più in prospettiva, del federalismo fiscale. Il nostro voto di astensione in prima lettura aveva proprio il senso di riportare un po' di realismo in una eccessiva enfasi che stava riguardando un testo che, pur introducendo alcune novità che tentavano di dare una soluzione all'ipertrofia legislativa della legge finanziaria, appariva a nostro giudizio, come è stato ricordato dal relatore Azzollini, dal relatore Azzollini, ancora generico, a contenuto prevalentemente centralista, sbilanciato a favore dell'Esecutivo e senza un efficace coordinamento con la recente legge di delega sul riassetto in senso federale dello Stato; tant'è che il lavoro importante sviluppato nell'altro ramo del Parlamento, con il contributo di numerose proposte emendative dell'opposizione, del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, ha portato ad una significativa riscrittura del testo. Il punto, allora, dal quale vogliamo ripartire nella discussione di oggi ha rappresentato e rappresenta un aspetto centrale di tutta la nostra iniziativa e ha trovato poi, a sottolineare anche che non vi era alcuna faziosità da parte nostra, una positiva rispondenza nelle scelte della maggioranza ed è il punto che a nostro giudizio riguarda il cuore dei problemi: in sostanza, il rapporto tra il Governo e il Parlamento. Anche dopo l'esperienza di questi ultimi anni, siamo convinti che se nelle procedure finanziarie e nelle regole contabili non si pone rimedio allo squilibrio strutturale che da un lato tuteli da un lato tuteli un'adeguata responsabilità del Governo e dall'altro fornisca al Parlamento validi strumenti di controllo, di indirizzo e ratifica, la finanza pubblica e la contabilità

prassi che vede accresciuto, con un arbitrio autarchico, il ruolo del Governo a discapito di quello delle Camere, mediante il ricorso da parte dell'Esecutivo a strumenti che noi consideriamo improponibili, quali manovre per decreto-legge e, prima ancora, finanziarie approvate con voto di fiducia su maxiemendamenti dell'Esecutivo, che all'assalto alla diligenza hanno sostituito improvvisazione, labilità legislativa e una sindrome da onnipotenza. c'è quindi l'esigenza di riequilibrare un processo decisionale chiaramente distorto, attribuendo al Parlamento un ruolo più incisivo sia in fase di rendicontazione e controllo (funzioni, queste, finora del tutto trascurate), sia in fase di concorso alla definizione degli obiettivi programmatici. Le modifiche apportate agli articoli 7 e 10 hanno fatto un passo in avanti - un piccolo passo in avanti - in questa direzione: il testo approvato dalla Camera precisa, infatti, che la decisione di finanza pubblica viene presentata alle Camere sotto forma di schema per le conseguenti deliberazioni parlamentari. pertanto, è che la Decisione di finanza pubblica diventi tale dopo il voto del Parlamento, ottenendo quindi un cambiamento significativo che consente di distinguere i diversi piani delle decisioni e di associarle poi a una complessiva visione del Governo. Un altro punto dolente che noi avevamo sottolineato è stato il raccordo tra il disegno di legge contabile e il provvedimento sul federalismo fiscale, dal momento che i due provvedimenti si sovrapponevano ed erano privi di un effettivo coordinamento. Noi avevamo chiesto che i provvedimenti contabili si adattassero alle novità invalse, con un occhio alle esigenze di impronta federalista e con l'altro a quelle di far di far collaborare tutte le amministrazioni all'obiettivo dell'unità economica della Repubblica, eliminando quindi qualsiasi rischio di strabismo legislativo. La questione di un'armonizzazione tra i sistemi contabili delle varie amministrazioni, non solo formale, ma sostanziale, è certamente per noi una premessa primaria di qualsiasi buona gestione di bilancio e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Nel nuovo testo, l'articolo 2, comma 6, inserisce pertanto principi nell'ambito della delega per l'attuazione del federalismo; l'articolo 10, comma 2, stabilisce che venga riportato il contenuto del Patto di convergenza e del Patto di stabilità nella decisione di finanza pubblica; l'articolo 11, comma 3, lettera *b)*, apporta una specifica di non interferenza su tributi, addizionali e compartecipazioni delle Regioni.

i governi di Regioni ed enti locali dovranno avviare per tempo la concertazione sul Patto di convergenza affinché lo schema di questo possa essere pronto nel momento in cui il Governo dovrà avviare una seconda fase di concertazione sul Patto di stabilità. modo, per noi resta aperta una contraddizione, in quanto nel testo della legge di contabilità non si prevede l'intesa in materia di Patto di stabilità, come previsto invece nella legge 5 maggio n. 42. Signora Presidente, in passato si partiva spesso da una debolezza strutturale: l'enorme ampliamento delle dimensioni e dei contenuti normativi della legge finanziaria si è spesso manifestato anche attraverso la prassi di affiancare uno o più decreti-legge collegati, che hanno reso ancora più complessi e confusi i procedimenti parlamentari, sia di indirizzo che di controllo.

cadendo nell'illusione di poter mettere un freno alla spesa con strumenti di intervento e di contenimento automatico e trasversale attraverso i cosiddetti tagli lineari, non selettivi, delle dotazioni di bilancio. Una migliore conoscenza e trasparenza sono d'altra parte il contrappeso necessario per assicurare al Parlamento, a fronte della maggiore flessibilità gestionale del Governo, un esercizio più efficace dei poteri di indirizzo e controllo. Un aspetto per noi rilevante della riforma è pertanto il rafforzamento di tutti i processi che concorrono al miglioramento del monitoraggio, del controllo e della valutazione dei conti pubblici. Certo, si deve fare ancora di più. comma 4 dell'articolo 11 prevede che al disegno di legge di stabilità venga allegato un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra. In questo senso, la banca dati prevista dall'articolo 14, alimentata da tutte le amministrazioni pubbliche, rappresenta sicuramente un passo in avanti nella direzione del maggior coinvolgimento delle autonomie, così come la riscrittura dell'articolo 40 sull'analisi e sulla valutazione della spesa, per rendere efficace il processo di programmazione ed efficiente l'allocazione delle risorse, istituzionalizza la prassi della cosiddetta *Spending* *Review*.

che rischierebbero però - lo dico al rappresentante del Governo - di restare teoria e astrazione se non venissero messe in atto tutte le garanzie affinché questi processi interagiscano tra di loro e si sviluppino in modo integrato. Restano comunque alcuni margini di possibile miglioramento e questioni aperte che richiedono da parte nostra una vigile attenzione.

che hanno l'obiettivo di dare garanzia di certezza rispetto alle attività intraprese dal Governo e i risultati conseguiti nella lotta all'evasione fiscale, nonché sull'efficacia delle misure adottate per contrastare la diffusione e il crescente fenomeno dell'evasione fiscale. Nell'ordine del giorno è inoltre rafforzata la previsione che il Ministro dell'economia trasmetta ogni anno al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive, con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali spostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici. Non a caso, il procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato relativo al 2008 ha ribadito che esistono degli annosi problemi tuttora irrisolti della lotta all'evasione che riguardano l'indebolimento dell'apparato sanzionatorio, l'indebolimento giuridico degli studi di settore e il *deficit* di conoscenza e trasparenza che caratterizzano l'approccio all'evasione. Sono dichiarazioni della Corte dei conti, quindi non strumentali, faziose o appartenenti ad una visione di parte. La stessa Corte dei conti poi, nella sua relazione depositata a gennaio, ha evidenziato, signor Vice Ministro, forti perplessità sulle iniziative intraprese dal Governo in materia di semplificazione e lotta all'evasione,

che, in attuazione della legge n. 296 del 2006, ha provveduto a presentare con ritardo alle Camere una relazione che era semplicemente una sommatoria di dati forniti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate.

mediante la previsione, signor Vice Ministro, di quattro diverse disposizioni di delega conferite dal Governo: entro un anno, decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili; sempre entro un anno, decreti legislativi per il potenziamento dell'attività di analisi; entro due anni, decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura di bilancio; entro tre anni, poi, il passaggio alla redazione del bilancio di sola cassa. evidente a tutti che la valutazione finale della portata e delle novità contenute in questa riforma e il successo reale della loro attuazione dipenderà molto dall'attuazione di queste importanti deleghe conferite al Governo. Il nostro impegno potrà esplicarsi con un atteggiamento positivo e propositivo, purché si vada nella direzione di una maggiore trasparenza e funzionalità di quella che noi vogliamo definire una riforma che punta a una moderna democrazia di bilancio.

alcune considerazioni su quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi in seguito all'applicazione di una così importante riforma, anche e soprattutto alla luce dell'accelerazione che la crisi sta imponendo a tutto il sistema di finanza pubblica non solo italiano ma anche degli altri Paesi. Faccio un esempio: è notizia di oggi che l'indice di povertà elaborato dell'agenzia di *rating* Moody's riporta un dato abbastanza particolare, cioè che l'Italia

sorge spontanea una perplessità. Eppure è una considerazione non di poco conto perché questo indice viene calcolato sommando il tasso di *deficit* pubblico e il tasso di disoccupazione.

il PIL è solo in via molto mediata oggetto delle scelte del Parlamento e del Governo. La stessa

quanto di tale incremento è discrezionale (cioè qual è la possibilità di agire), come vengono spese le risorse e quali sono gli indicatori di efficienza ed efficacia nell'uso di queste risorse.

nel momento in cui il problema si sposta non tanto sulla speranza che ci sia una crescita da rincorrere, eventualmente con un aumento di imposte (se non basta la crescita per finanziare un aumento di spesa), quanto

programmazione economica e bilancio: già oggi, nelle competenze delle Commissioni bilancio, sia della Camera che del Senato, vi è un'azione che non è solo quella di analisi della finanziaria e di analisi della copertura, ma anche di analisi di come vengono spesi questi 80 miliardi di euro. Tenendo conto che più della metà è in capo ai Ministeri centrali, a maggior ragione è competenza delle Commissioni economiche, sia della Camera che del Senato, operare un profondo controllo di gestione, di verifica e anche, avendo a disposizione degli indicatori extracontabili, di creazione di indicatori che consentano di capire come vengono spesi i denari dei contribuenti.

Questi 80 miliardi di euro provengono per metà da un'operazione di bilancio e per metà dallo scudo fiscale, che è un'azione *una tantum.*

segnalato all'Aula come sia assolutamente impensabile continuare, come se nulla fosse, ad incrementare la spesa pubblica, sperando che il buon Dio faccia aumentare le entrate con un non meglio specificato effetto di aumento della domanda mondiale. Ora, è evidente a tutti che noi non possiamo più permetterci questo livello di spesa, come è evidente a tutti che dobbiamo razionalizzare la spesa e cercare di combattere l'evasione fiscale.

In quest'ottica, a nostro avviso, è assolutamente evidente che si arriverà a una specializzazione delle competenze delle Commissioni bilancio di Camera e Senato,

è evidente che, implicitamente e necessariamente, si produrrà una specializzazione e una differenziazione delle competenze delle funzioni delle due Commissioni bilancio e anche dei due Servizi

e con l'auspicio che si arrivi a un compimento pieno, con i decreti attuativi, affinché tale riforma diventi davvero lo strumento agile e snello per consentire al Parlamento di ragionare più sul controllo

*(PD)*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, l'impianto di questa riforma è il frutto di un dibattito risalente negli anni, ed è il frutto di apporti tecnici e politici di grande qualità: una discussione all'altezza del compito che il Parlamento si è dato nell'esprimere

ai colleghi, al relatore, al collega Morando ed a molti altri che hanno dato un apporto importante nel definire la qualità di questo testo legislativo: un testo, appunto, frutto di una cooperazione vera tra maggioranza ed opposizione, che ha portato, almeno in prima lettura, ad una sua scrittura condivisa. Ciò mi porta ad una prima considerazione di carattere generale: quando si vogliono fare riforme utili al Paese

La seconda considerazione che volevo fare riguarda l'enfasi che si è voluta dare nel corso di questi mesi, riecheggiata anche nella discussione di questa importante riforma, all'organizzazione della scansione temporale della sessione di bilancio ed ai contenuti degli strumenti

DPEF, al 15 settembre (quindi in un tempo che consente di registrare meglio gli andamenti dell'economia e della finanza pubblica ed il contenuto della legge di stabilità e della legge di bilancio), nonché dei collegati entro il 15 febbraio:

Io certo non sono nostalgico - nessuno di noi credo lo sia - delle vecchie leggi finanziarie, ma l'esperienza di quest'anno, a partire dal decreto n. 112 del 2008, ci dimostra che così non è; ce lo dimostra la legge finanziaria così com'è venuta a configurarsi alla Camera in questi giorni, per contenuto, ampiezza e per superamento anche di quei limiti che erano stati indicati con il citato decreto n. 112, ma soprattutto ce lo dimostra la qualità della produzione legislativa di questi mesi e dell'ultimo anno,

di quegli interventi, non siamo molto lontani dalle vecchie leggi finanziarie che abbiamo visto negli anni. Così come credo sia stata eccessivamente enfatizzata - ho avuto modo di sottolinearlo durante la prima lettura - la necessità di eliminare dalla legge di stabilità, dalla vecchia legge finanziaria, le norme

ci fa correre il rischio che possa venir meno una visione unitaria delle politiche di sviluppo e della politica economica, che prima in qualche modo veniva garantita.

è tanto più elevato, se si tiene conto del fatto che non si è voluto attribuire, come noi avevamo proposto, un carattere cogente ai tempi di approvazione dei collegati alla legge finanziaria che contenessero

contabilistica vigente), ma ciò che è ancora più importante è il costume politico e la Costituzione materiale, nonché la concezione dei rapporti tra Governo e Parlamento, soprattutto in questa delicata fase storica,

Prima vi era la possibilità per il Parlamento di incidere in misura maggiore nel rapporto con il Governo e di modificare, se del caso, l'impostazione di politica economica

le indicazioni programmatiche inserite in questo provvedimento viene tendenzialmente spostato verso il Governo. Il Parlamento, allora, come esce da questa riforma? Questa è la riflessione che vorrei proporre,

Il collega Mascitelli poco fa ha richiamato la modifica che è stata apportata alla Camera, in base alla quale si prevede ora espressamente che la Decisione di finanza pubblica debba essere quella risultante dall'approvazione dei

È stato detto con dovizia di particolari e con argomenti pregevoli, che non voglio in alcun modo riprendere nel merito, che la soppressione della struttura unica di supporto tecnico a disposizione del Parlamento e della Commissione parlamentare per la trasparenza dei conti pubblici costituisce una grave ed inaccettabile mutilazione dei poteri effettivi del Parlamento. Il nostro consenso si basava su un assetto di questo tipo: da un lato, l'accrescimento non solo

chi detiene storicamente e ancora oggi il potere vero di determinare o meno decisioni di finanza pubblica, a volte importanti, o decisioni che comunque impattano sulla finanza pubblica? C'è una sola fonte informativa, a disposizione del Governo e del Parlamento; a volte infatti, secondo l'esperienza che abbiamo potuto

troppo limitati, eccessivamente contenuti. Vogliamo citare qualche esempio di attualità? Noi da qualche anno, con un dibattito molto avanzato discutiamo della famosa introduzione della cedolare secca sui canoni di locazione; da anni, e quest'anno più degli altri, abbiamo registrato la condivisione unanime del Parlamento su questa misura, che è necessaria, è utile al Paese e nel medio e lungo periodo sarà utile anche alla finanza pubblica. Ebbene, da anni la Ragioneria generale dello Stato dice che non si può fare, non si può fare, perché costa troppo, perché non è vero che gli effetti virtuosi si vedranno dal primo o dal secondo anno, forse dal terzo. Il Parlamento è pertanto impedito dall'assumere una decisione così importante, destinata ad avere riflessi sul mercato immobiliare, sul bene casa,

Il Parlamento non è posto nelle condizioni di assumere una decisione consapevole e di munirsi a sua volta di uno strumento informativo che gli consenta di assumere una decisione consapevole.

ottenere finalmente la ragionevole durata del processo, la maggioranza, con l'assenso del Governo, sostiene che far durare i processi non più sei anni o dieci ma due anni non costa niente. È possibile una cosa del genere? Abbiamo chiesto al Governo di fornire una Relazione tecnica: com'è possibile che uno dei più grandi problemi italiani,

far durare i processi poco, se si vuole ottenere un processo rapido occorre investire di più, in mezzi, personale, organizzazione: occorrono le risorse. Eppure, il Governo e la maggioranza hanno provato a convincerci che così non è. Quindi, noi di quali strumenti disponiamo? Eppure, lei, presidente Baldassarri, ci ha intrattenuto (e noi abbiamo prestato attenzione alle sue proposte) sul fatto che sarebbe possibile con la legge finanziaria tagliare la spesa corrente dello Stato di 37 miliardi di euro (o 40, non ricordo), e ha configurato

Noi eravamo e siamo convinti che tagliare 37 miliardi di euro non è possibile, ma può darsi che avesse ragione il presidente Baldassarri, del bilancio dello Stato si possano reperire risorse da destinare o orientare diversamente da quanto avviene oggi, senza smantellare

ragione quanti di noi ritengono che fare operazioni in quei termini quantitativi (non mi riferisco all'aspetto qualitativo), a occhio e croce non sia possibile? Non disponiamo di strumenti Ecco quindi che il tema che è stato posto dal collega Morando è di primaria importanza. Non è un aspetto marginale del dibattito in corso È in gioco il potere del Parlamento di essere informato sulle grandezze finanziarie, sull'impatto finanziario derivante dalle misure adottate, sugli andamenti di finanza pubblica, di disporre cioè di un'autonoma, autorevole fonte informativa, propria, sulla base della quale poter svolgere il lavoro che ci compete e in questo senso alimentare il contraddittorio ed il confronto con il Governo.

Questo è un problema politico di primo ordine, a mio avviso. Ecco perché insistiamo: insistiamo perché è ragionevole che si reintroducano quelle norme, perché le avete condivise e votate in prima lettura.

non uno, ma molti provvedimenti? Sulla base di che cosa ragioneremo con riferimento all'impatto sui territori, sulle Regioni, sui Comuni, sulle Province, sulla fiscalità generale? Sulla base di che cosa? Sulla base di dati che verranno partoriti non sappiamo dove o da chi, dati non riscontrabili? Insomma, gli argomenti sono molteplici per ritenere che se vogliamo fare per davvero una riforma condivisa, seria, che serva al Paese, e vogliamo farla, possiamo apportare qui i cambiamenti necessari a cui ci siamo riferiti e che sono oggetto dei nostri emendamenti, dei quali discuteremo. Se lo faremo, avremo fatto una cosa importante per il Paese; altrimenti, avremo fatto una mezza riforma che, a mio modo di vedere, avrà necessità di ulteriori interventi e, comunque, non sarà quella di cui il Paese aveva ed ha bisogno. *(Applausi

Non posso non far mie le parole pronunziate dal Capo dello Stato sull'aggressione subita nel pomeriggio di domenica scorsa dal Presidente del Consiglio, al quale rinnovo ogni augurio di pronta guarigione. Non solo, quindi, «la più ferma condanna del grave e inconsulto gesto di aggressione nei confronti del Presidente del Consiglio», ma anche «il più netto, rinnovato ogni contrasto politico e istituzionale sia ricondotto entro limiti di responsabile autocontrollo e di civile confronto, prevenendo e stroncando ogni impulso e spirale di violenza». Ho già avuto modo di esprimere personalmente al Presidente del Consiglio, unendomi a quanto detto dal Capo dello Stato, la mia sincera solidarietà. Ma sono certo di interpretare l'animo di tutto il Senato nel rivolgere un appello accorato a tutte le forze politiche e sociali affinché, concordemente, si interrompa questa spirale di violenza ed aggressività verbale nei confronti degli avversari che, come la storia insegna, può con facilità trasformarsi in aggressività e violenza fisica. Il nostro Paese ha già conosciuto stagioni di odio che tanto dolore hanno portato ai nostri concittadini e tante divisioni laceranti tra le forze politiche e nel corpo sociale. Facciamo tutti uno sforzo concorde per evitare che nuovamente i fantasmi della violenza civile - con incoscienza da qualcuno evocati - tornino ad aggirarsi nella vita quotidiana del nostro Paese. Gli avversari politici siano tali, in un confronto magari anche aspro e duro, ma non divengano mai nemici da abbattere e distruggere con la violenza. E l'unica via per spezzare questo rincorrersi ed accelerarsi di incomunicabilità, di accuse, di violenze verbali (e ormai purtroppo non soltanto verbali) è quella di fermarsi, discutere e confrontarsi su quel terreno delle riforme del sistema politico ed istituzionale che poche settimane fa ha visto maggioranza e opposizione parlare finalmente, qui in Senato, un linguaggio comune. *(Applausi).* Ha facoltà

lo sdegno mio personale e di tutto il Governo per la gravissima aggressione di cui il Presidente del Consiglio è rimasto vittima nella serata di domenica a Milano. A lui va la mia incondizionata solidarietà e vicinanza, con l'augurio che possa al più presto tornare a svolgere la sua preziosa attività alla guida del Governo. L'eccezionale gravità dell'accaduto richiede una puntuale ricostruzione dei fatti. Nel pomeriggio di domenica scorsa, in occasione dell'apertura della campagna di tesseramento, il Popolo della Libertà ha organizzato una manifestazione in piazza Duomo a Milano, in un'area che, soprattutto in vista delle prossime festività natalizie, è particolarmente frequentata. L'iniziativa si è svolta in una zona retrostante il Duomo e contigua a corso Vittorio Emanuele, dove era stato allestito il palco per gli oratori, e prevedeva la presenza di numerose autorità, tra cui il sindaco di Milano Letizia Moratti, il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, numerosi Ministri e il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 10.000 persone; essa è iniziata intorno alle ore 17,15 e il Presidente del Consiglio è arrivato sul posto intorno alle ore 17,40. Fin dall'inizio le forze di polizia impiegate nel servizio di ordine pubblico hanno rilevato la presenza in piazza di un centinaio di persone che contestavano la manifestazione e il Governo. I contestatori sono stati subito fronteggiati dai reparti di polizia schierati sul posto, che li hanno fatti arretrare sino in piazza Duomo, angolo via Santa Radegonda. L'intervento dei reparti scongiurava ogni contatto tra i contestatori e i manifestanti, evitando ulteriori scontri e più gravi turbative allo svolgimento della manifestazione. Un altro gruppo di quattro o cinque persone, anch'esse contestatori, si è posizionato sotto il palco all'esterno delle transenne, innalzando bandiere del Popolo della Libertà: all'arrivo del Presidente del Consiglio, dopo aver abbandonato le bandiere, il gruppo ha tentato di srotolare a favore delle telecamere uno striscione con una scritta ingiuriosa nei confronti del Presidente del Consiglio. Anche tale tentativo veniva scongiurato dal pronto intervento degli operatori di polizia presenti, che riuscivano ad evitare che la provocazione potesse degenerare in episodi più gravi. Il Presidente del Consiglio, dopo aver chiamato sul palco i Ministri presenti, il sindaco di Milano e il presidente della Regione Lombardia, chiudeva la manifestazione e, intorno alle ore 18,35, raggiungeva l'area immediatamente retrostante il palco, ove erano state disposte ad attenderlo le autovetture del dispositivo di sicurezza. A questo punto il Presidente, prima di ripartire, ha deciso di fermarsi per rispondere alle domande di alcuni giornalisti e per salutare i numerosi cittadini posizionati dietro le transenne predisposte per recintare la zona retrostante il palco. È proprio in questa occasione che, alle spalle dei giornalisti e delle persone che salutavano il Presidente, confusa tra la folla, una persona - successivamente identificata come Massimo Tartaglia, di 42 anni, residente a Cesano Boscone con un'azione improvvisa lanciava contro il presidente Berlusconi un oggetto in alabastro riproducente il Duomo di Milano, da lui comprato in precedenza in un chiosco della piazza. Il presidente Berlusconi veniva colpito al volto, tra la bocca e il naso, riportando gravi ferite e un vistoso sanguinamento. Portato immediatamente presso l'ospedale San Raffaele per le necessarie medicazioni, è stato successivamente ricoverato con una prognosi di 25 giorni per ferite lacero-contuse al labbro superiore e distacco della porzione più distale della spina nasale ed osso mascellare di sinistra. L'aggressore è stato immediatamente bloccato da un operatore del servizio di sicurezza e dal personale del locale commissariato di polizia e sottratto al tentativo di aggressione di altre persone presenti sul posto. Accompagnato in questura, subito dopo il fermo, è stato interrogato dal pubblico ministero Armando Spataro, che ne ha disposto l'arresto per il reato di lesioni volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale della parte offesa e dalla premeditazione. Il Tartaglia - come da lui stesso dichiarato in sede di interrogatorio - si trovava in prossimità del luogo della manifestazione già dalle ore 11 del 13 dicembre, proprio in preparazione del suo folle gesto. In particolare, la premeditazione risulta provata anche dalla circostanza che l'aggressore è stato trovato in possesso di una bomboletta spray al peperoncino e di altri oggetti contundenti, astrattamente idonei a ledere le persone, tra cui un crocifisso in materiale resinoso. Il Tartaglia ha dichiarato di non appartenere a gruppi politici organizzati né di frequentare centri sociali, ma di aver agito da solo, spinto dalla rabbia che da tempo covava dentro di sé nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Dai primi accertamenti è risultato che l'aggressore - celibe, incensurato e destinatario unicamente di un provvedimento di revoca della patente di guida per sopravvenuta mancanza dei requisiti - è da molti anni in cura per problemi psichici di tipo paranoico e ha problemi di lavoro, nonché grosse difficoltà relazionali con i genitori. Al momento sono ancora in corso le indagini da parte della polizia giudiziaria e il Tartaglia è stato condotto presso il carcere di San Vittore. La gravità dell'episodio mi ha indotto a incontrare personalmente nella mattinata di ieri, presso la prefettura di Milano, i rappresentanti delle forze dell'ordine. Ho voluto subito effettuare un'accurata ricostruzione dei fatti per verificare se il sistema di gestione dell'ordine pubblico durante la manifestazione fosse stato predisposto ed attuato secondo le regole che devono essere rispettate in casi del genere. La mia convinzione è che ciò sia avvenuto e che nessun rilievo possa essere mosso ai responsabili milanesi dell'ordine pubblico. I dispositivi attuati hanno anzi consentito di sventare, come ho prima ricordato, un tentativo di violenta contestazione al Presidente del Consiglio proprio sotto il palco. Ricordo che, in occasione di ogni visita o impegno pubblico del Presidente del Consiglio, vengono preventivamente effettuati sopralluoghi da parte di personale della questura in stretta collaborazione con personale dell'AISI (l'Agenzia per la sicurezza interna), a cui compete direttamente la responsabilità della sicurezza e della protezione istituzionale del Presidente del Consiglio dei ministri. Vengono altresì disposti minuziosi servizi di bonifica preventiva sui percorsi e sui luoghi interessati, nonché specifici servizi di osservazione e riservata vigilanza da parte del personale della Digos. I luoghi che saranno visitati dal Presidente del Consiglio vengono, già dalla giornata precedente, debitamente sorvegliati mediante l'istituzione di servizi di vigilanza fissa. Vengono inoltre allertati tutti i servizi di vigilanza in corso ed attivate tutte le fonti informative al fine di individuare preventivamente, anche mediante il monitoraggio della rete Internet, eventuali iniziative di contestazione e protesta, al fine di predisporre le opportune contromisure. Inoltre, la sicurezza personale curata dal personale dell'AISI è sempre supportata, a largo raggio, anche da personale della questura che opera in abiti civili a loro stretto contatto. Il compito delle forze dell'ordine in situazioni come quella attuale è di particolare delicatezza e complessità: coniugare in ogni momento la doverosa garanzia della libertà di manifestazione del pensiero di chiunque con l'altrettanto doverosa esigenza di tutelare la sicurezza e l'incolumità dei dei rappresentanti delle istituzioni del Paese, al pari di tutti i cittadini. È proprio la ricerca di questo delicato punto di equilibrio che contraddistingue l'impegno delle forze dell'ordine in circostanze come quelle vissute domenica pomeriggio in piazza del Duomo a Milano. Ma l'asprezza dei toni che la dialettica politica ha recentemente assunto e, più in particolare, la progressiva, crescente campagna contro la persona del Presidente del Consiglio dei ministri, che in molti casi travalica le regole del legittimo confronto democratico, finisce per innescare spesso una pericolosa spirale emulativa. Dopo la gravissima aggressione di domenica è ripresa la proliferazione su alcuni *social network* come «Facebook» di gruppi che inneggiano all'aggressione del Premier che, come è già accaduto nel recente passato, incitano alla violenza nei confronti di Berlusconi. L'autorità giudiziaria è già stata attivata al riguardo, ma stiamo valutando ogni possibile iniziativa legislativa per contrastare la diffusione di messaggi che integrano la fattispecie di veri e propri reati, quali l'istigazione a delinquere e l'apologia di reato. Finora i tentativi in sede parlamentare di introdurre nel nostro ordinamento norme efficaci in tal senso hanno dovuto segnare il passo rispetto alle difficoltà di individuare interventi mirati a colpire solo i messaggi violenti, senza coinvolgere la generalità degli utenti dei *social network* che utilizzano l'opportunità delle moderne tecnologie della rete per fini assolutamente leciti. Ricorderete che proprio il Senato ha recentemente discusso e approvato una norma, poi cancellata dalla Camera, che introduceva la possibilità per il Ministro dell'interno di intervenire in questi casi.

vengono commessi dei reati sul *web* e ad intervenire. Vogliamo dare - ed è questo il senso della norma che sto studiando - un potere effettivo alla magistratura, che credo sia l'organo più competente in materia, per decidere non semplicemente se ci sono dei messaggi violenti, ma se ci sono dei messaggi che integrano dei veri e propri reati per interromperne la commissione. Sto pertanto valutando soluzioni normative - che intendo sottoporre alla discussione del prossimo Consiglio dei ministri - che siano appunto compatibili con queste esigenze, grazie anche all'esperienza operativa maturata dal servizio della Polizia postale e delle comunicazioni, già proficuamente attivo nel monitoraggio della rete per l'individuazione dei siti e delle pagine *web* che inneggiano alla violenza. È proprio grazie ai proficui contatti tra il servizio della Polizia postale e delle comunicazioni e la società statunitense proprietaria di «Facebook» che è stato possibile intervenire nello scorso mese di ottobre per rimuovere i messaggi che, anche in quell'occasione, istigavano alla violenza contro il Presidente del Consiglio. Sono infine in corso approfondimenti di livello tecnico per verificare, anche qui, la possibilità di iniziative legislative per contrastare più efficacemente gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni pubbliche, in un quadro di compatibilità con l'ordinamento vigente, sulla falsariga di quanto già avviene per combattere la violenza negli stadi. Il Governo nella sua collegialità e il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, si sentono attivamente impegnati a garantire la sicurezza di tutti i cittadini e di tutti i rappresentanti istituzionali, a partire dalle più alte cariche dello Stato, nell'interesse del regolare svolgimento della vita democratica del Paese e in particolare della imminente campagna elettorale per le prossime elezioni regionali e amministrative. È auspicabile, al riguardo, che gli stessi temi della sicurezza delle più alte cariche istituzionali e dei cittadini non rappresentino un ulteriore motivo di dannosa e strumentale polemica politica. È proprio per questo che occorre raccogliere l'invito del Presidente della Repubblica e quello fatto pochi minuti fa dal Presidente del Senato affinché, pur nella diversità delle varie posizioni politiche, si fermi la pericolosa esasperazione della polemica politica e si torni al più presto ad un normale, civile confronto tra le diverse parti politiche e le diverse istituzioni.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei esprimere, a nome del Gruppo Misto, in tutte le sue componenti, i sentimenti di piena solidarietà e di vicinanza, umana e politica, al presidente del Consiglio Silvio Berlusconi per la gravissima aggressione di cui è stato vittima domenica sera in piazza del Duomo a Milano. Un'aggressione che palesa drammaticamente il clima di tensione che da mesi sta contagiando il Paese come un virus al quale bisogna porre rimedio prima che degeneri e raggiunga livelli che possano mettere a rischio la civile convivenza nel nostro Paese. Ringrazio anche il Ministro dell'interno per l'informativa resa in quest'Aula e per aver sottolineato la capacità delle forze dell'ordine di garantire la sicurezza dei cittadini nel pieno rispetto dei principi fondamentali di uno Stato democratico. Tuttavia, il volto insanguinato del Presidente del Consiglio è segno, comunque, di una violenza che mai deve appartenere alla democrazia. In questo clima, che non esitiamo a definire di vera e propria istigazione all'odio, avvertiamo l'esigenza di una responsabile riflessione della politica che deve riguardare tutti, indistintamente. Anche perché in Italia, si sa, la solidarietà non regge all'usura delle ventiquattr'ore. E non vorrei che, nei prossimi giorni che verranno, si ritornasse a quello scontro politico che ha costituito l'*humus* nel quale è maturato il vile attacco contro il Capo del Governo. Dobbiamo tutti abbassare i toni: lo dico ai colleghi dell'opposizione e ai colleghi della maggioranza, perché c'è un'aria troppo avvelenata, dove la mancanza di serenità è del tutto evidente. In questi mesi c'è stata un'*escalation*, fin troppo emotiva, che ormai pervade ogni ambito della politica, ogni comunità, dalle piccole amministrazioni alle grandi Regioni, dove la polemica politica ormai è vittima di questa tensione che vede arbitrariamente la divisione tra buoni e cattivi e la denigrazione degli avversari-nemici senza avere alcun riguardo per il valore reale di ogni singola persona, della comunità e dei cittadini, ridotti a meri spettatori di così riprovevoli comportamenti. Tutto ciò deve cessare immediatamente. Dovremmo raccogliere tutti l'invito che viene dalle parole del Capo dello Stato, quando dice che «viviamo un'esasperazione pericolosa della polemica politica che bisogna fermare» per ritornare «a un normale e civile confronto tra le forze politiche e le istituzioni. Non ha senso che gli uni accusino gli altri per il clima che si è creato». Anche per questo, penso che il gesto del segretario del maggiore partito dell'opposizione, di recarsi in visita all'ospedale San Raffaele dall'onorevole Berlusconi, sia stato un segnale importante dal quale bisogna ripartire. un gesto che vale più di mille parole e che respinge con i fatti le farneticazioni di quanti vorrebbero continuare a masticare odio e rancore perché è l'unico modo che conoscono di concepire l'opposizione politica a un Governo e al suo *leader*. Chiunque ha il diritto di esprimere le proprie idee, anche con forza, senza che questo significhi essere demiurghi di ambiguità dalle quali possono nascere oscure violenze. Vorrei anche dire che la cifra di quanto avvenuto domenica a Milano risiede proprio nella deriva che vede la politica divisa in fazioni contrapposte, una sorta di eterna guerra tra il bene e il male, dove il confronto, la dialettica e persino la legittima contrapposizione politica sono spesso sostituite da risentimenti e da una cruda quanto gratuita violenza verbale alimentata da determinate e ben individuabili testate giornalistiche. Facciamo tesoro dunque di questa brutta pagina della democrazia italiana per riflettere tutti insieme sulla pericolosa deriva che ha preso la dialettica politica nel nostro Paese. Si torni ad affrontare con serietà i temi e i problemi che attanagliano la vita quotidiana degli italiani. Si abbandonino il livore e il preconcetto ostile per trovare, invece, un comune più alto senso del nostro dovere parlamentare. Dimostriamo con i fatti che le condanne, le espressioni di solidarietà, le giuste affermazioni negative dell'accaduto sono trasformate in atti concreti a salvaguardia di un bene superiore, qual è - appunto - la democrazia. Con questo, nel ribadire gli auguri al presidente Berlusconi per una pronta guarigione e un immediato ritorno alla guida del Paese, auspichiamo che il senso di responsabilità prevalga sulla strumentalizzazione fine a se stessa, da qualsiasi parte essa provenga, e che si inverino nei fatti le parole, da tutti condivise, del Capo dello Stato.

degli estremismi di destra e di sinistra), l'Italia debba trovare l'unitarietà di tutte le forze politiche del Parlamento nella condanna nei confronti di un atto che poteva compromettere la vita del Presidente del Consiglio. sentimenti che ci sentiamo di esprimere con molta sincerità sono una solidarietà piena al Presidente del Consiglio e una vicinanza umana all'onorevole Silvio Berlusconi, a cui auguriamo una pronta guarigione. Tante parole sono state spese su questa brutta e drammatica vicenda che, attraverso il grave attentato al presidente Berlusconi, ha anche arrecato un danno gravissimo all'immagine internazionale del nostro Paese, proprio per l'evidenza mediatica dei fatti. Troppe parole, a volte inutili, sono state purtroppo pronunciate anche in Parlamento, anche alla Camera dei deputati questa mattina, e sui giornali. Le responsabilità, l'odio, i mandanti morali: un dibattito stucchevole e preoccupante, tutto teso ad aggirare la questione principale che con molta saggezza e con grande semplicità il Presidente della Repubblica ha evidenziato e che lei ha ripreso nel suo intervento introduttivo. Cioè l'esigenza di isolare i violenti, i falchi, quelli che nei vari schieramenti, a destra e a sinistra, lucrano sullo scontro e non sul confronto politico, che affidano il proprio futuro e le proprie fortune politiche e giornalistiche (mi riferisco anche ad autorevoli giornali della destra italiana) alla alla necessità di alzare sempre e comunque il tono del dibattito usando ad arte un linguaggio violento, provocatorio, che serve solo ad alimentare lo stato d'animo delle proprie tifoserie. Ecco, quello che noi dobbiamo fare oggi, il segnale che dobbiamo dare tutti insieme è proprio quello di isolare le tifoserie, tifoserie, i falchi, coloro i quali lucrano dalla incompatibilità e dall'assenza di dialogo le proprie fortune e il proprio futuro politico. La terza considerazione, signor Presidente, riguarda la questione della sicurezza del Premier. Noi abbiamo ascoltato le parole del Ministro dell'interno e non potevano che rassicurarci dal punto di vista della funzionalità generale della sicurezza che riguarda il Premier come, ovviamente, tutte le alte cariche dello Stato. dello Stato. Però ci sono due problemi che devono essere affrontati. Il primo è che la sicurezza del Presidente del Consiglio è un bene indisponibile.

gesti di emulazione e quindi la circostanza che il Presidente del Consiglio, per sua scelta, ritenga di dover sempre e comunque incontrare le folle non è più possibile.

sono in vigore in maniera efficace dal 2006. In questo contesto, signor Presidente, ci associamo alle sue parole e a quelle del Capo dello Stato, convinti però che la necessità di un confronto sereno debba partire da fatti, gesti e atti concreti. Noi per primi in questi anni, in questa in questa legislatura, ne abbiamo fatti tanti e continueremo a farli perché riteniamo che oggi l'elemento più importante sia il confronto: il confronto scevro da ogni forma di violenza, anche verbale, che può dare la sensazione e l'illusione di una percentuale di consenso in più a questa o a quella forza politica, ma che alla fine produce quei risultati che tutti noi contestiamo e che siamo costretti oggi a condannare.

Se io fossi il pubblico ministero di quel processo, contesterei all'indagato e arrestato

che possa giustificare un atto criminale. Sono motivi abietti perché è abietta quella politica.

perché così facendo faremmo rientrare nella politica ciò che mai, per nessuna ragione, può appartenere alla politica. Vi siete chiesti perché i cittadini, tuttora, in un sondaggio in corso, esprimono un giudizio secondo cui, dopo il grave episodio di violenza, il clima della politica nel nostro Paese è peggiorato?

alla politica, ossia alla sua incapacità di sottrarsi ai tentativi speculativi? Noi dobbiamo con forza e unità dire a tutti che la violenza non è uno strumento della democrazia e dire ai cittadini che la politica è fatta anche di contraddizioni dure, anche di espressioni forti,

e ai fatti del Governo e della maggioranza. Ci confrontiamo e scontriamo su temi obiettivamente forti, importanti per il nostro Paese e per i cittadini. dei Valori non ci faremo condizionare dalle speculazioni e, nel rispetto della democrazia, continueremo senza esitazione a svolgere il ruolo di opposizione decisa alle proposte o ai fatti che dovessimo giudicare dannosi per il Paese e di opposizione costruttiva attraverso le nostre proposte in Parlamento e le attività nelle sedi proprie della democrazia. Non accetteremo mai che qualcuno ci dica come si fa l'opposizione. Così come riteniamo che nessuno possa dire che, ad esempio, il Presidente della Camera abbia armato la mano del folle avendo dichiarato che il presidente Berlusconi da monarca assoluto, insofferente ad alcune regole del nostro sistema democratico. Non lo pensiamo e faremmo un torto alla democrazia se qualcuno lo pensasse o lo dicesse. Dobbiamo dimostrare maturità democratica. Noi esprimiamo, come Italia dei Valori, il nostro augurio di pronta guarigione al presidente Silvio Berlusconi. Vogliamo poi esprimere l'ulteriore augurio che quest'Aula solenne trovi un momento di sintesi superiore, perché tutti insieme, convinti e decisi, si possa dire sì alla democrazia, sì alla politica, no alla violenza!

una carovana di carta e un carosello di immagini hanno raccontato la drammatica aggressione al Presidente del Consiglio, al quale vanno tutta la nostra solidarietà, la nostra sentimenti che la Lega Nord nutre senza ipocrisia, con in lealtà ed entusiasmo. Voglio provare a pescare nell'universo di parole spese in questi giorni tre concetti che mi paiono fondamentali. Il primo si riferisce alle dichiarazioni del ministro dell'interno Maroni, allorquando egli ha affermato che Silvio Berlusconi poteva essere ucciso. Se è vero che l'aggressore è una mente fragile,

origina la considerazione che l'agguato si sia consumato in un clima fortemente conflittuale e, soprattutto, in una temperie alla quale il termine odio non è estraneo. In secondo luogo, pur pur condividendo l'invito ad abbassare i toni, rispetto alla violenza verbale non mi sento di sottoscrivere un principio di equidistanza tra centrodestra e centrosinistra. Se si vogliono evitare ipocrisie, almeno oggi, affermiamo con chiarezza che nessuno mai, come il nostro Presidente del Consiglio, è stato fatto oggetto di attacchi concentrici che non possono non far lievitare il germe della violenza.

questo lo schema che, anche oggi, ho letto sui tradizionali giornali dei cecchini del Premier. Il terzo punto riguarda le preoccupazione che si ricreino terribili climi già conosciuti nel nostro Paese. I messaggi su «Facebook» che sono stati ricordati, inneggianti all'eroe Tartaglia, sono un segnale gravissimo, perché indicano che l'odio è in atto e che ogni parola spesa male può essere benzina per i più esagitati ed irresponsabili. Questo episodio non deve essere isolato dal contesto sociale, né tanto meno sottovalutato. C'è chi ha decretato il crepuscolo di Berlusconi e chi ha provveduto a mettere in atto una sorta di giustizia Il Parlamento deve tornare a dare l'esempio, ridando alle parole il loro significato e alle contrapposizioni il loro peso. Soprattutto, in una fase nella quale parte del Paese è in sofferenza, sappiamo che quelle condizioni sociali possono essere strumentalizzate dai meno avveduti, da coloro che confondono l'antagonismo con l'odio e che non esiterebbero a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di sopraffare, se non sopprimere, l'avversario. Concludo, signor Presidente, dicendo che occorre dunque stare all'erta, frequentare ciascuno di noi la categoria della responsabilità, sapendo che il clima può essere surriscaldato anche in previsione delle prossime consultazioni elettorali. Auguri di cuore al presidente Berlusconi e al nostro Paese, che ne ha tanto bisogno.

voglio formulare al presidente Berlusconi, a nome del mio Gruppo naturalmente, e a nome mio personale, non solo la nostra solidarietà ma anche gli auguri di un ristabilimento pronto e di una una possibilità di riacquistare una serenità che in questi giorni, come ci è sembrato di capire, è stata perduta, non solo in ragione delle ferite e quindi del danno fisico che ha riportato, ma anche di un'inquietudine psicologica in ordine ad un sentimento molto profondo di ingiustizia, che ha manifestato con ripetute affermazioni circa il clima di odio che nei suoi confronti si è sviluppato, secondo l'apprezzamento del Presidente. Non ho da qualificare altrimenti che come gesto criminale l'attacco rivolto nei confronti del presidente Berlusconi e il mio intervento, colleghi, piuttosto che piuttosto che guardare soltanto alle reazioni che si sono susseguite in questi giorni, di cui i colleghi ci hanno parlato e di cui stamattina si è parlato alla Camera e che in questi giorni hanno affollato le pagine dei giornali e le immagini delle riprese televisive, vuole descrivere quello che penso essere un momento un po' complicato, difficile e comunque delicato della vita della Repubblica. Penso che noi tutti, e mi riferisco ovviamente anche ai colleghi della maggioranza, siamo nel dibattito di questi giorni come dirigenti politici, e come dirigenti politici adulti e, ci auguriamo reciprocamente, anche come dirigenti politici responsabili. Ciascuno di noi sa bene, molto più di quanto non lo possa sapere il cittadino che accende la TV o che legge i giornali, quale possa essere la conseguenza anche immediata di ogni nostro gesto e di ogni nostra parola. Siamo degli esperti del simbolo e anche della comunicazione, come dicono gli esperti di linguaggio subliminale. Per questo credo, e penso così di leggere e rappresentare l'interesse e la volontà del mio Gruppo e del mio partito, che può talvolta anche essere e qui e ora secondo me è necessario - prescindere dalle voci che si alzano, come accaduto stamattina alla Camera, e trovare in sé la misura del momento e del proprio comportamento. La nostra misura, signor Presidente, colleghi, ministro Maroni, è quella adeguata alla seconda forza politica del Paese, al più grande partito di opposizione di un'Italia che certo ha le sue difficoltà ma che è una delle più importanti democrazie europee. Non staremo quindi alla tentazione di una discussione che ancora oggi rischia di ad avvitarsi nella spirale dell'aggressività e della reciproca delegittimazione tra maggioranza e opposizione. Noi rappresentiamo più di 12 milioni di italiani e ci facciamo carico, perché ci tocca, di questi cittadini ma anche di tutti coloro i quali non ci hanno votato ma che pretendono di vivere in un Paese in cui lo scontro politico, duro e intransigente quando occorre, non degeneri mai in tensioni che tocchino la saldezza delle istituzioni e che facciano sentire qualcuno di questi cittadini in balia di eventi imprevedibili e rischiosi. Noi siamo una grande forza tranquilla. Ovviamente, neanche per un attimo rinunceremo alle nostre idee e alle nostre proposte, ma abbiamo le spalle abbastanza grandi per respingere il rischio di ogni provocazione. Faremo il nostro lavoro senza cedimenti e rappresentando ogni giorno - ci auguriamo - la possibilità di discutere rendendoci utili al Paese. Lo dico pensando alla mozione sulle riforme che abbiamo discusso in quest'Aula la settimana scorsa, su nostra iniziativa, e lo dico pensando anche al modo con cui si è ritenuto, invece, di andare all'approvazione della finanziaria alla Camera, perché pensiamo che questo sia il nostro atteggiamento e la misura dello stesso, e il nostro auspicio è che, anche con queste dichiarazioni di voto, in questo senso possa

- siamo ancora convinti che per recuperare la misura di questa nuova relazione politica tra le diverse forze non ci sia la necessità di nessuna legge nuova o eccezionale. Lei ha mostrato anche stasera in un passaggio, che pure era complesso, di sapere, come ciascuno di noi, quanto fragile sia la libertà di manifestazione del pensiero e quanto sia denso di rischi ogni intervento legislativo che incida o possa incidere su di essa. Stiamo attenti a non cercare altrove quello che invece sta nella nostra capacità di trovare la misura virtuosa di esercitare il massimo della conflittualità politica nel massimo rispetto delle regole democratiche. Nessuno di noi ha una scorciatoia; a ciascuno di noi tocca fare un pezzo e nessuno di noi può pensare di non avere niente da correggere, niente da ripensare, niente da riflettere.

Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, signori del Governo, stasera intervengo in vece del nostro Capogruppo, presidente Maurizio Gasparri, al quale un grave lutto ha impedito di essere presente e per il quale gli rinnovo la vicinanza mia e di tutti i senatori del Popolo della Libertà

lei ci ha confermato che i fatti di cui parliamo oggi in quest'Aula non possono essere derubricati ad un seppur grave incidente di percorso, dovuto alla miscela tra una mente instabile e un generalizzato clima di odio di cui tutti saremmo corresponsabili e che dovremmo tutti impegnarci a superare. Signor Ministro, è in atto da mesi un'operazione concentrica di criminalizzazione ai danni del Presidente del Consiglio, con attori e comprimari. Con la stessa franchezza dobbiamo rilevare che vi è stato uno spartiacque in questa prima parte della legislatura. Un momento che ha segnato un'involuzione nella vita del Paese e a seguito del quale la campagna d'odio contro Berlusconi e l'azione combinata di forze para-eversive ha compiuto un evidente salto di qualità. È una constatazione, non un giudizio di valore. Mi riferisco alla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato il «lodo Alfano». Una decisione che, a scanso di equivoci, rispettiamo fino in fondo, ma in merito alla quale non possiamo fare a meno di ribadire il nostro giudizio negativo, sul piano tecnico e sul piano politico. Perché in un solo colpo essa ha spazzato via un seppur imperfetto tentativo di ripristinare l'equilibrio fra giustizia e politica pensato dai Padri costituenti e infrantosi nel 1993. Ha inoltre eluso il principio di leale collaborazione fra le istituzioni, contraddicendo un pronunciamento precedente e traendo in inganno il legislatore (circostanza sulla quale i tanti colleghi dell'opposizione, che più di chi parla dicono di tenere alla centralità del Parlamento, farebbero forse bene a riflettere). *(Applausi Soprattutto, nei fatti e al di là delle intenzioni, ha dato forza a quanti intendono mettere in discussione la legittimità del potere democratico consacrato dalla volontà del popolo. Signor Presidente, negli ultimi mesi è stata infranta la diga del confronto civile. È stato possibile che il Premier, il Presidente del Consiglio di questo Paese, fosse additato come corresponsabile delle stragi di mafia; che fosse chiamato in causa in mondovisione da un sedicente pentito, del quale per carità di patria evitiamo in questa sede di ripetere il *curriculum*; un sedicente pentito ammesso in un pubblico dibattimento senza uno straccio di prova ma dopo un lungo accreditamento preventivo a mezzo stampa. È stato possibile che la storia politica scritta negli ultimi 15 anni dalla maggioranza degli italiani fosse riletta come una sorta di "romanzo criminale", nei tribunali e sulla televisione di Stato, nelle piazze e sui giornali. Colleghi, per noi questo è il momento di mettere da parte le ipocrisie: noi ascoltiamo l'appello del presidente Napolitano e faremo la nostra parte, fino in fondo. questo non esonera nessuno di noi da un'analisi obiettiva del passato recente; e non autorizza nessuno a mettere tutti sullo stesso piano Perché da parte di questa maggioranza campagne d'odio *contra personam* non se ne sono mai viste, e mai saremmo rimasti alleati di chi se ne fosse reso responsabile. Insomma, ben venga un richiamo comune, purché nessuno pensi di potersi mondare la coscienza con un generico «chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato». Proprio la capacità di graduare le responsabilità ci porta in queste ore a cogliere significative differenze all'interno dell'opposizione. Senatore Li Gotti, abbiamo colto anche gli accenti del suo discorso, e non la prenda come una provocazione ma come una constatazione: è sembrato quasi un intervento in dissenso rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal leader del suo partito. atto che i Comitati di liberazione nazionale sono finiti ancora prima di nascere; soprattutto, apprezziamo il gesto compiuto dall'onorevole Bersani, il più semplice e per questo il più sincero. Allora rilanciamo ai nostri avversari la sfida delle riforme che in questa stessa Aula ci ha visto compiere un passo significativo. Diciamo loro: rendiamo l'Italia una democrazia compiuta, circostanza che presuppone legittimazione reciproca e la messa al bando di qualsiasi tentazione di conquistare il potere attraverso scorciatoie giudiziarie. Facciamo in modo, signor Presidente, che la residua speranza che tutto ciò sia possibile non resti sepolta in piazza Duomo a Milano, sotto una coltre di odio e di menzogna.

Purtroppo, però, a causa di una ristrutturazione, e non quindi di una situazione di crisi, intende licenziare i dipendenti dell'azienda che operano nella sede e delle politiche sociali, anche se l'azienda non intende adottare la cassa integrazione per i dipendenti, di interessarsi di questa ristrutturazione e quindi di porre in essere una soluzione di cassa integrazione al fine di valutare la suddetta ipotesi di ristrutturazione. Credo che, di fronte ad una condizione di ristrutturazione e non di crisi, sia doveroso da parte del Governo intervenire in questo senso. È inusuale, ma non sempre le situazioni inusuali sono situazioni impossibili. Riteniamo che, proprio di fronte ad una situazione di non crisi, sia doveroso che il Governo intervenga in tal senso.

Ieri si è svolto un ulteriore incontro in prefettura con tutti i sindaci della provincia di Napoli, che hanno espresso una solidarietà molto ampia per questa realtà produttiva, tra le più importanti del Mezzogiorno, con il vescovo di Nola

e non è stata neanche confermata l'anticipazione della cassa integrazione speciale per il prossimo anno. Vi è di più. Circa 140 giovani operai altamente specializzati, che avevano un contratto a termine con quello stabilimento, il 31 dicembre vedranno conclusa la loro esperienza lavorativa. Sono giovani monoreddito altamente professionalizzati. Il dramma sociale si aggiunge dunque alla grave crisi e al dramma dei lavoratori.

- come ho detto prima - una delle più importanti e significative realtà produttive del Mezzogiorno vedrà la chiusura.